Grazie,

«La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguente condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 1, comma 11, siano aggiunte in fine le seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14, articolo 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108." Il parere è altresì reso nel presupposto che, in relazione all'articolo 3, comma 5, non si determinino effetti peggiorativi rispetto agli andamenti tendenziali della spesa, alla luce della prassi amministrativa già applicata nel quadro della legislazione vigente. In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo sulle proposte 1,1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10 2.2, fermo restando tuttavia che, ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tutti i restanti. Il parere è quindi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.8, 1.9, 3.7 (testo 2), 3.201, 3.202, 3.203, 3.205, 3.5, 3.6 (testo 2) e 3.10. Esprime poi parere non ostativo sulla proposta 3.200, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la riammissione in servizio sia subordinata alla perdita di indennità alternative e che venga soppressa la clausola di copertura.

3.200 (testo 2) e 3.250 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 3.250 e parere di semplice contrarietà

l'evidente inammissibilità di alcuni emendamenti e quindi per sollecitarne la declaratoria da parte sua. In particolare, mi riferisco

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G101, esprimo parere contrario, anche perché parte da premesse che si sono rivelate assolutamente inesatte, come quella secondo cui il presidente Obama avrebbe recentemente affermato la necessità di una progressiva riduzione dei militari impegnati al fine di mettere in atto una *exit strategy:* è esattamente il contrario di quello che sta accadendo.

Per quanto concerne l'ordine del giorno G104, mi rimetto al Governo. Ho peraltro forti dubbi, perché nel momento in cui

Il Governo esprime parere contrario in ragione del linguaggio molto critico sull'azione del Governo e sul ruolo dell'attuale diplomazia, che è utilizzato sia nelle premesse che nel dispositivo e che il Governo non giudica accettabile.

a: coinvolgere le rappresentanze militari nella discussione sulle materie di competenza in analogia a quanto avviene per le parti sociali; valutare la possibilità di aprire la discussione su un sistema di previdenza complementare per il personale militare; valutare la possibilità di aprire una discussione sulle possibili misure atte a superare la condizione di precariato del personale di truppa; avviare la riforma della rappresentanza militare; consentire una ampia discussione degli organismi di rappresentanza di ogni livello con la base rappresentata sui contenuti della riforma.

dal 2003 le missioni internazionali di pace hanno sempre avuto nel bilancio dello Stato un Fondo ad esse dedicato. Ovviamente, questo fondo è stato puntualmente e periodicamente rimpinguato a seconda delle decisioni politiche assunte in sede internazionale, che hanno determinato obblighi per il nostro Paese.

per la parte di suo interesse e, contemporaneamente, l'occasione per fare una riflessione più generale sull'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali. Ora, nella finanziaria per il 2010 questo Fondo è scomparso. Abbiamo sollevato, prima in sede di discussione in Commissione poi con quest'ordine del giorno, l'attenzione sul significato politico che la scomparsa di questo Fondo rischia di assumere, soprattutto tenendo conto del fatto che, come ricordato ieri

Ora, immaginare che questa situazione possa essere trattata volta per volta, a discrezione totale del Ministro dell'economia per quanto attiene al suo finanziamento, pone due problemi il primo è che, in tal modo, trasmettiamo all'esterno del nostro Paese il senso della provvisorietà su come trattiamo la presenza delle nostre missioni nel mondo;

Come ho già detto, se fino a qualche giorno fa poteva esserci il dubbio, ad esempio nel caso dell'Afghanistan, che la presenza della NATO avrebbe potuto subire una decisione di totale ridimensionamento in virtù della posizione americana,

entra in una fase profondamente diversa e che, se fino a qualche giorno fa esistevano dubbi che potesse essere mantenuto l'impegno così come è stato sinora

Per queste ragioni, insistiamo sul voto favorevole sull'ordine del giorno G100. Confidiamo che la discussione sulla finanziaria che si sta svolgendo nell'altro ramo del Parlamento, anche alla luce degli eventi che si sono determinati in queste ultime ore, induca il Governo a modificare il suo atteggiamento e a ristabilire il Fondo per le missioni internazionali nel bilancio, per dare a queste

e deve continuare ad avere soprattutto nel migliorare e rafforzare il ruolo dell'Italia nell'ambito delle missioni internazionali, se è vero, come è stato ricordato, che siamo uno

Per queste ragioni, il nostro Gruppo chiede di votare, non accetta le richieste di modifica e non capisce l'atteggiamento del Governo, che ha espresso parere contrario sull'ordine del giorno

il Governo può difficilmente accettare un ordine del giorno che nella parte iniziale del dispositivo reca un giudizio negativo sull'azione del Governo e questo penso sia facile da comprendere da parte sia della maggioranza che dell'opposizione. Ma vi è qualcosa in più. Il dispositivo, alla fine, impegna il Governo a sviluppare nelle opportune sedi ed organismi internazionali un'azione diplomatica e politica, cosa che il Governo sviluppa tutti giorni, davanti agli occhi di tutti quelli che sono stati i contatti con la NATO, con l'ONU e con i Paesi partner da parte del ministro Frattini, del ministro La Russa e del Presidente del Consiglio.

favorevole a che il nostro impegno all'estero si concretizzasse nel modo migliore possibile - di accettare una forma di finanziamento in divenire, che si confrontasse con le entrate dei conti pubblici, ma che ci desse in prospettiva, come ci ha dato quest'anno, la possibilità di arrivare ad un finanziamento del 40 per Queste sono le motivazioni, da una parte comprensibili e, dall'altra parte, di ordine strategico, guardando al risultato e non soltanto alla teoria, che mi portano a dare parere contrario sull'ordine del giorno G100.

Crediamo, infatti, che sulla cooperazione allo sviluppo finalizzata al sostegno dei progetti di pace, di stabilizzazione, nonché allo sminamento dei territori interessati in passato dai conflitti armati sia necessaria una maggiore programmazione Gli obiettivi stessi della stabilizzazione sono realizzabili solo con azioni di lungo periodo e con progetti pluriennali.

che procedere con un finanziamento di soli due mesi fosse assolutamente limitante. È mia convinzione infatti che non sia corretto legare imprescindibilmente a livello temporale - se non altro - questo genere di interventi internazionali (ossia, la cooperazione allo sviluppo)

al 30 giugno del 2010. In particolare, l'emendamento 1.1 prolunga fino al 30 giugno 2010, anziché al 31 dicembre 2009, il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Somalia, Sudan, nonché agli interventi di sminamento umanitario anche in altre zone e territori di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, indicando la cifra da stanziare per questi scopi per i primi sei mesi del 2010. Riteniamo che questo emendamento vada

Senatore Di Giovan Paolo, come lei ben saprà, la portata di un ordine del giorno è di gran lunga inferiore alla portata di un emendamento e ci sono molti precedenti di emendamenti

1.100,

Come avevamo già dichiarato durante il dibattito nelle Commissioni riunite, uno dei motivi per cui in effetti, almeno per quanto mi riguarda, su alcuni di questi emendamenti non ci poteva essere convergenza è che si vanno a cercare i finanziamenti necessari con una pratica diffusa durante la cosiddetta prima Repubblica (che, però, ahinoi, non è mai finita): si andavano cioè ad aumentare le tasse sulle sigarette, detta in soldoni. Sappiamo che la creatività del Governo Berlusconi, complice anche buona parte dell'opposizione, è riuscita a creare invece un altro meccanismo per finanziare alcuni trattati internazionali, cioè l'aumento dell'addizionale IRES. Al centro di molti degli interventi del senatore Pedica in Commissione vi è stata

multinazionali, molto spesso controllate dal Governo, in parte anche in modo abbastanza rilevante. Quindi, si vanno a fare commesse di vario genere a genere a controllate o a amici di amici. Come si è fatto in occasione del trattato di amicizia Italia-Libia, quando si sono recuperati i soldi tassando coloro che poi avrebbero beneficiato delle commesse di costruzione di strade, case, ponti, aeroporti

All'articolo 2 si prevede infatti la sostituzione del comma 1, contenente la proroga della missione relativa all'Afghanistan, ipotizzando di porre una proroga fino al 28 febbraio 2010, in luogo del 31 dicembre 2009, comprensiva dei costi per il rientro definitivo dei nostri contingenti. Abbiamo ritenuto che un lasso di due mesi per procedere ad un definitivo rientro sia un tempo indicativo e di massima assolutamente assolutamente ragionevole per organizzare un disimpegno concordato con i partner internazionali, in sede ONU e NATO, che che permetta un passaggio di responsabilità nelle mani di altri Paesi membri che partecipano alla missione, o ancor meglio, nella responsabilità delle forze afgane locali, ormai assolutamente legittimate dalla nuova presidenza Karzai alla quale tutti, dagli Usa alla Francia e all'Inghilterra - lo ha ribadito anche Obama questa notte - stanno chiedendo di assumere il diretto controllo dell'ordine e della sicurezza nel Paese. Quella contenuta nell'emendamento non è una fuga o un frettoloso rompete le righe, ma la richiesta di concordare multilateralmente un disimpegno graduale che si concluda entro il 28 febbraio. Per permettere ciò abbiamo stabilito una copertura finanziaria adeguata, ossia a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009 la spesa di euro 84.481.907, nonché l'ulteriore spesa di euro 115.518.093 per l'anno 2010, comprensiva dei costi per il rientro dei contingenti, per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan denominate *International Security Assistance Force*. Signora Presidente, così non posso continuare il mio intervento. Lei ha più volte ripreso l'Aula: le chiedo cortesemente di continuare a farlo e di non usare due pesi e due misure.

nella sua acritica posizione di conservazione dello *status quo* della missione in Afghanistan. Una missione di guerra e non di pace; una missione senza fondi economici sufficienti per sostenerla; una missione contraria allo spirito della Costituzione; una missione che i cittadini, e l'Italia dei Valori con loro, non vogliono più. Con responsabilità mi rivolgo soprattutto ai colleghi del Partito Democratico, dell'UDC e anche della Lega, le cui posizioni sono tutt'altro che in linea con quelle oltranziste del Popolo prima di votare su questo emendamento e assumetevene la piena responsabilità. Noi, con coraggio e responsabilità, lo abbiamo fatto e continueremo a farlo.

e a tutti i senatori dell'Italia dei Valori di riflettere prima di compiere un atto così grave come la

di grande portata, tanto da risultare inidoneo al servizio militare incondizionato, in attività operative, addestrative o nello svolgimento del servizio la possibilità di essere richiamato in servizio *sine die*. È una forma di attenzione che ritengo assolutamente necessaria, che si rivolge ad un certo numero di militari; si tratta di tutti quelli che ricordiamo ogni volta che si verifica un incidente in Afghanistan o in altri teatri,

perché, magari, non tutti i nostri colleghi hanno avuto l'opportunità di approfondire la questione delle norme contenute in questo provvedimento e, forse, non hanno avuto il tempo necessario per ponderare quanto è stato incluso non soltanto nella fase di dibattito che ha visto la presentazione di una serie di emendamenti, alcuni fortunatamente dichiarati improponibili, ma anche nella preparazione della misura stessa. Il comma 7 recita: «Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze

attenzione - «è prorogato fino al 30 luglio 2011». Oggi siamo al 2 dicembre 2009: quindi, un anno e mezzo di proroga dei vertici delle rappresentanze militari, COCER e COBAR. Il deputato radicale nel Gruppo del Partito Democratico Maurizio Turco ha portato avanti per tre settimane uno sciopero della fame per porre due questioni:

in una fase politica come la nostra, dove addirittura si è voluto creare un ulteriore giorno in memoria dei caduti civili e militari su teatri di guerra che vedono la nostra presenza in missioni internazionali, noi, per riconoscere lo straordinario lavoro dei nostri militari, arriviamo a non far esprimere loro la preferenza relativamente a chi li deve rappresentare. Ieri, il sottosegretario Cossiga si è ampiamente dilungato su una serie di questioni che non avevano a che fare con il dibattito in Aula, riservando solo due brevi risposte

noi ci saremmo ovviamente dichiarati contrari. Ripeto: qui si vuole congelare per un anno e mezzo il diritto codificato e sancito dalla Costituzione di trattare i militari come tutti i cittadini.

Condividiamo le preoccupazioni testé espresse dal collega Perduca, nel senso che questo diritto costituzionalmente garantito rappresenta non soltanto una modalità di partecipazione alla vita democratica, ma anche un ambito di intervento rispetto al quale le varie forze politiche sono impegnate addirittura per un miglioramento. Tuttavia, non ci sentiamo di condividere le affermazioni del collega Perduca allorché afferma che l'approvazione di questa proposta determinerebbe un congelamento delle libertà e delle garanzie del mondo militare.

ogni possibile azione legata agli opportuni veicoli legislativi per approdare ad una nuova normativa sulla rappresentanza.

in ordine al ruolo delle Forze armate sono tali da non poter più essere ristorate dalla previsione attuale. Pertanto, ciò che viene presentato come un modo per intralciare l'espressione del parere e delle sensibilità delle Forze armate in verità altro non è se non uno sforzo per impostare in modo migliore il lavoro.

tralascio di leggere il comma 7 dell'articolo 3 perché è stato già letto dal collega Perduca. L'emendamento 3.14 è soppressivo del suddetto comma perché esso impedisce ai cittadini militari di eleggere nuovi rappresentanti alla scadenza naturale del mandato, cioè nella primavera del prossimo anno. Siamo in disaccordo perché di fatto si viene meno al fondamentale principio di democraticità degli organismi, sancito dall'articolo 18 della legge n. e si impedisce per un tempo troppo lungo agli aventi diritto, specialmente dopo la previsione del mandato quadriennale rinnovabile, di premiare o respingere con l'espressione di voto le idee e le posizioni assunte dai rappresentanti uscenti. Pur comprendendo la motivazione fornita dal Governo nella relazione illustrativa, secondo cui, a giustificare l'urgenza di tale intervento normativo, vi sarebbe una procedura per il rinnovo dei suddetti organi troppo lunga e complessa che potrebbe non concludersi in tempo, riteniamo più opportuno pensare ad una norma che provveda allo snellimento della procedura di elezione, anziché autorizzarne lo slittamento.

Grazie degli equivoci rispetto alla materia su cui detto emendamento inciderebbe. Si tratta in realtà non di fondi unici per la sicurezza né di altre materie che erroneamente sono state da qualcuno

incrementati *una tantum* con altre disposizioni), ma le procedure attivate per l'attribuzione degli stessi si sono rivelate sostanzialmente inefficaci. Con l'emendamento in questione si propone pertanto di prevedere che tale attribuzione venga determinata attraverso un decreto interministeriale (che vede quindi il

Siccome i nostri sono lavori pubblici - credo, peraltro, trasmessi in diretta in questo momento da Radio radicale - le affermazioni del sottosegretario Crosetto sono gravissime. Non so se lui sia stato eletto o no, ma l'esempio che ha portato non calza neanche un po': sarebbe come dire che noi, al terzo anno di legislatura, decidiamo che la nostra legislatura dura sette anni e mezzo. Questo era l'esempio che doveva fare il Sottosegretario! Allo stesso tempo, visto e considerato che queste sono le analisi del Governo, mi meraviglio dell'ottimismo del Gruppo del Partito Democratico, che dà fiducia alla maggioranza e al Governo perché si possa arrivare ad una revisione revisione profonda del sistema con cui vengono elette le rappresentanze dei nostri militari. Ho ricordato poco fa lo sciopero della fame dell'onorevole Turco, radicale nel Gruppo del PD alla Camera, che ha interrotto la sua

la stessa: contrariamente a quanto molto leggermente affermato poco fa dal rappresentante del Governo, si va a sospendere un diritto civile di persone che vestono una uniforme.

Ricordo anche che a 45 giorni delle elezioni europee di quest'anno si è deciso - tutti concordi, tranne alcuni rappresentanti del Movimento per le autonomie e i radicali - di modificare una legge elettorale. Quindi, quando si sa che ci sono delle scadenze certe che sicuramente presentano diverse problematiche e si sa, allo stesso tempo, che si è dalla politica chiamati a porre rimedio a questo tipo di problemi - che, lo ripeto, non sono problemi di legge ma politici - si trova anche il tempo (magari la notte) di modificare i regolamenti. Perché questa volta non lo si vuole fare? Sicuramente ci sono dei giochi che tutti conoscono e che magari non ci interessa affrontare in questa fase di dibattito, giochi tra esclusi o persone che pretendono di andare a rappresentarne altre. tutto ciò va contro la nostra Costituzione che, tra l'altro, è molto chiara relativamente al limite con cui le nostre forze militari possono essere impiegate. Se da una parte noi continuiamo a rispettare la norma che ci impedisce di partecipare a guerre, ma esclusivamente a missioni internazionali sancite da decisioni assunte da organi regionali come l'Unione europea, la NATO e le Nazioni Unite, dall'altra dovremmo stare attenti, allo stesso tempo, ad onorare il servizio dei nostri militari, concedendo loro il pieno godimento di tutti i diritti civili e politici. Quindi, almeno sull'ordine del giorno

proposta per l'introduzione di un codice penale militare adeguato alla realtà delle missioni internazionali, cosa che evidentemente costituisce ulteriore rafforzamento di molti inviti che il Parlamento nei suoi due rami già negli anni passati con maggioranze diverse aveva sempre rivolto. E, in effetti, il Governo, come preannunciato dal ministro La Russa qualche mese fa, è in procinto - è questione, da quel che risulta, di pochi giorni - di presentare all'approvazione del Consiglio dei ministri un disegno di legge delega per la emanazione di un codice penale militare riferito specificamente alle missioni internazionali.

troverà - come siamo certi - la sua approvazione, successivamente il Governo potrà emanare, sulla base della delega, il codice penale militare delle missioni, ferma restando l'ulteriore necessità di provvedere comunque alla In questi ultimi mesi - ma la questione era risalente - si sono evidenziate delle urgenze relative alla disciplina penale, e quindi alla protezione dei nostri militari impegnati nelle missioni. In particolare, si sono evidenziate delle preoccupazioni in ordine - come si ricorderà - alla vicenda del sequestro operato dalla magistratura dei mezzi offesi in alcune operazioni ai fini dell'accertamento delle responsabilità, attraverso meccanismi (che non sono in questo senso processuali)

più accelerata, che sia quindi compatibile con le necessità di reimpiego di quei mezzi dopo che siano stati svolti gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria in Italia. Proprio per questo è prevista anche l'introduzione della possibilità di notifica di alcuni di questi provvedimenti per via telematica, cosa che attualmente non è prevista, e che ha costituito, per esempio, il burocratico accidente che, al di là della volontà dei magistrati inquirenti, ha in effetti ritardato il il reimpiego di quei mezzi dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. In sostanza, quindi, con l'emendamento 4.200 si propone di introdurre un meccanismo che preveda tempi certi e nello stesso tempo rapidi (10 giorni prorogabili con un motivato ulteriore provvedimento del pubblico ministero) e che quindi sia possibile, anche attraverso la la notifica dei provvedimenti per via telematica, risolvere e superare quei problemi che si sono evidenziati proprio nei tempi recenti. Con l'emendamento 4.201, invece, si chiede l'introduzione, nel merito,

per la missione dell'Afghanistan, in aderenza a quanto in precedenza era stato modificato da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati e poi confermato dal Senato ancora nella scorsa legislatura, con il quale era stata reintrodotta l'applicazione del codice penale militare di pace al posto del codice penale militare di guerra, che in precedenza era applicato per le missioni in Iraq e in Afghanistan. Dicevo che non esiste nella disciplina vigente una causa di giustificazione specifica perché, ovviamente, quelle che sono previste dal codice di pace non presuppongono che vi possano essere attività anche di difesa e di reazione ad attacchi

che, conformemente alle regole di ingaggio, al diritto internazionale, alle disposizioni impartite, siano costretti a far uso della forza, e in particolare a far uso delle armi. Quindi, l'emendamento che si propone in qualche modo anticiperebbe una disposizione che sarà poi compiutamente e stabilmente introdotta, qualora ovviamente il Parlamento ne approvi il contenuto, con il codice penale delle missioni internazionali e che fa riferimento al fatto che, appunto, non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2 (cioè di quelle oggetto della proroga con il presente

il reato di eccesso colposo qualora i limiti dei comportamenti qui indicati siano stati ecceduti per colpa e quindi non con dolo. Credo sia importante, proprio per le situazioni più recenti che si sono che si sono ulteriormente ripetute, in particolare nello scenario afgano, che il Parlamento accordi una tutela chiara, precisa e puntuale ai nostri militari che sono impegnati costantemente in questa difficile opera

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,

intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole e per esprimere pubblicamente un apprezzamento nei confronti del relatore

tant'è che la 5a Commissione, che prima aveva ritenuto di non dover dare il proprio parere favorevole, ha trovato poi il modo per reperire i fondi necessari. Speriamo che questo atteggiamento di libertà

rilevo questa assenza importante, nonostante sia chiaro che la discussione di oggi sia di fondamentale importanza e di enorme delicatezza; nonostante ci siano state fuori dal Senato manifestazioni contro questo provvedimento; nonostante questa notte il Presidente degli Stati Uniti ci abbia detto quale strategia intende attuare in Afghanistan, ovverosia l'invio di altri 30.000 uomini, con la prevedibile conseguenza che questo voto sul rifinanziamento delle missioni per solo due mesi assume un significato molto ampio: l'avallo o meno della politica estera italiana in Afghanistan per i prossimi anni. Nonostante tutto ciò, il Presidente del Consiglio si sente molto probabilmente in pace con la sua coscienza, perché non ha ritenuto un dovere intervenire questa mattina, forse perché con i mezzi propri di un dittatore ha considerato sufficiente l'averci annunciato, tramite un comunicato stampa redatto il 25 novembre, che anche l'Italia contribuirà con maggiori uomini - si parla di 1.500 - alla missione ISAF. Benissimo: ne prendiamo atto. allora la mia dichiarazione di voto come la inizierebbe il mio presidente Di Pietro: «Signor Presidente del Consiglio che non c'è», la posizione dell'Italia dei Valori sul provvedimento è dolorosamente attenta alla situazione dei militari, alle finalità di pace delle missioni e alla ormai mutata natura della missione in Afghanistan, regolata dall'articolo 2, comma 1, del decreto. Certo, oltre all'articolo 2, comma 1, esistono diverse criticità che non abbiamo esitato a rilevare (e che avete ignorato bocciando i nostri emendamenti). Innanzitutto, l'incongruenza di finanziare per soli due mesi la cooperazione allo sviluppo, quando questa si articola su progetti pluriennali - appunto, di «sviluppo» - che certo non può essere conseguito e valutato in soli 60 giorni. Ed è per questo che abbiamo proposto di aumentare il termine, finanziario ma quindi anche operativo, fino al 30 giugno 2010. In secondo luogo la soppressione, all'articolo 3, comma 7, delle consultazioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti delle Forze armate nel COCER. Un atto che mina il principio democratico della rappresentanza elettiva e lascia presumere accordi fra i rappresentanti parasindacali e il Governo. Ma non mento se affermo che, al di là di questi importanti rilievi, è la nostra presenza militare in Afghanistan che condiziona la nostra posizione ed il nostro voto. Colleghi, la guerra in Afghanistan è iniziata ormai da 8 anni. Dall'invasione del 2001 che ha rimosso i talebani dal Governo, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno ripetutamente optato verso soluzioni rapide e non sostenibili sul lungo periodo. È stata una guerra lampo, a cui è seguita però una lenta e perdurante sconfitta - direi - i cui effetti concreti appaiono in tutta la loro drammaticità adesso. I numeri, a volte, sono molto indicativi. Lasciate che ve li illustri. Dopo otto anni d'occupazione in Afghanistan da parte di forze internazionali guidate dagli Stati Uniti, i talebani che si dovevano sconfiggere sono presenti sul 97 per cento del territorio. Dall'invasione nel 2001 dell'Afghanistan ad oggi la guerra ha causato la perdita di circa 43.000 vite umane. Secondo dati di fonte internazionale, al settembre di quest'anno i civili uccisi in Afghanistan erano 7.589, i soldati afgani morti in combattimento 11.000, 6.000 i soldati e gli agenti di polizia, 25.000 i guerriglieri, 1.400 i soldati USA e NATO, 21 i soldati italiani; i feriti, tra militari e civili, oltre 53.000. Il 2009 risulta essere inoltre l'anno più sanguinoso per le forze internazionali dall'inizio del conflitto. Chi si stringe intorno al dolore dei familiari dovrebbe sapere che le due missioni di *peace-keeping* in Iraq e Afghanistan hanno prodotto 753.399 morti. «Missioni di pace»,

perché quella indicata da Obama sembra più un'utopia che una mossa finale: subito l'invio di 30.000 soldati e fra tre anni l'inizio del loro ritiro. realtà. sappiamo benissimo che sul "subito" la politica può decidere, ma sul futuro di qui a tre anni a nessuno è dato disporre. considerato poi, in aggiunta agli allarmanti dati che vi illustro, un ulteriore fattore per valutare il successo o il fallimento di una politica estera: la percezione che la popolazione locale ha delle forze straniere. L'annuncio che il ballottaggio delle elezioni presidenziali non avrebbe avuto più luogo ha rafforzato la sensazione nel popolo afgano di un sostanziale fallimento della democrazia, sia per colpe endogene all'amministrazione di Karzai, che per responsabilità europee e americane, in quanto la frettolosa benedizione che i Paesi NATO hanno dato a un Presidente che non è stato eletto da una maggioranza e con un Governo corrotto è apparsa come una sconfitta di quel sogno di democrazia che avevamo promesso agli afgani. Al cuore del fallimento nel costruire solide istituzioni non c'è tuttavia il numero insufficiente di uomini inviati dalle forze multinazionali, non il numero inadeguato dei cannoni piazzati sui nostri Mangusta, né quante bombe potevano esser sganciate in più per soffocare i talebani.

si possa fare non con la forza delle armi, ma con tutti quegli altri strumenti politici, economici e diplomatici che la comunità internazionale, e l'Italia, ha a disposizione. Proprio perché pensiamo che una soluzione al *dossier* Afghanistan non si trovi con il solo confronto militare, l'Italia dei Valori considera una netta contraddizione osservare che se l'Italia è il terzo Paese europeo per impegno militare nell'area, è invece il quindicesimo su tutti gli altri aspetti civili e di cooperazione. Non è mai chiaro quanto costi davvero una spedizione militare, ma per approssimazione nel 2008 sarebbero stati spesi 349 milioni di euro, circa 29 al mese, mentre quest'anno la cifra potrebbe raggiungere i 40 milioni al mese. Soldi per armi, non per cibo, farmaci o libri! Cari colleghi, come possiamo poi non considerare le conseguenze internazionali della nuova strategia americana annunciata questa notte? È una dura strategia d'attacco, che comporterà altrettanto dure reazioni da parte dei talebani; una strategia che porrà le truppe americane di fronte a nuovi pericoli, che risulteranno ancora più alti per le truppe italiane, le quali operano negli stessi teatri di statunitensi, ma non hanno né regole d'ingaggio offensive, né l'equipaggiamento, né i mezzi militari e neppure l'addestramento d'attacco proprio dei *marines* per rispondere in sicurezza alla controffensiva talebana. A fronte di tale accresciuto pericolo, gli altri Paesi europei hanno risposto molto tiepidamente e tutti, già da mesi e più o meno apertamente, stanno pensando alla conversione degli sforzi armati in progetti di natura civile.

fatto da Obama, la Germania esprime una posizione attendista, in vista della conferenza che si terrà a Londra il prossimo 28 gennaio. Da Parigi è netto il no alla richiesta americana per 1.500 uomini In Gran Bretagna Brown ha suggerito l'esigenza di definire una *exit strategy* da tenersi entro il 2010. E la Polonia il 9 novembre scorso ha votato una mozione di ritiro delle truppe entro agosto 2010.

perché ignora l'opinione pubblica, le posizioni dell'opposizione parlamentare, ma anche - cari colleghi del PdL e della Lega - le posizioni della maggioranza parlamentare. E allora, senatori, non vi sentite mortificati nel vostro ruolo ad essere qua a discutere della proroga missioni per soli due mesi, fino a dicembre, mentre a palazzo Grazioli hanno già deciso quanti soldati in più e per quanti anni verranno inviati a Kabul? Io, francamente, m'indigno e lo stesso fa il mio partito. Anche perché la notizia che invieremo 1.500 soldati non è stata affiancata da un dibattito che chiarisca al Paese né la natura di tale incremento armato, né la finalità, né la modalità operativa, ed anche perché questo ulteriore sforzo militare ci costerà 300 milioni di euro l'anno, quando solo ieri l'ISTAT

Forse il piano di Berlusconi è quello di mandare quel 30 per cento di giovani disoccupati a combattere la guerra in Afghanistan per salvare capra e cavoli? Perdonate il mio ampio discorso, ma esso è volto a illustrare come la posizione dell'Italia dei Valori non voglia cavalcare il malcontento popolare sull'Afghanistan, ma sia seria e dolorosamente responsabile.

il coraggio di ricordarsi cosa scrissero i Padri costituenti nel 1946 quando introdussero l'articolo 11 nella Costituzione, oggi da voi dimenticato. Il coraggio di dire che se l'Italia non è fatta per fare la guerra può comunque mantenere alto il suo impegno internazionale con mezzi politici, economici e diplomatici, che sa usare meglio di quelli della forza bruta. Questo coraggio ci ha portato oggi a votare contro l'articolo 2 del decreto proroga missioni e ci porta e ci porta adesso ad astenerci sul provvedimento nel suo complesso. La «proroga missioni» è un'espressione che da oggi, con questo primo significativo e simbolico gesto dell'Italia dei Valori, noi rifiutiamo, perché è impossibile prorogare senza ripensamenti una missione quando tutto il contesto locale muta attorno e quando Obama ci dice che la nuova strategia sarà di massiccio attacco, a meno di non apparire ciechi, incapaci di pensare una politica estera per l'Italia e schiacciati sotto il ricatto degli altri Paesi europei e degli Stati Uniti. E non oso pensare che questa caparbia ottusità

che davvero sono di pace, rimane nel provvedimento questa cieca e, lo dico, anche cinica volontà di lasciare che i nostri soldati, partiti cinque anni fa per costruire la pace, si ritrovino oggi a combattere la guerra che non hanno mai voluto. Con questo voto auspico che anche i colleghi ed il Governo compiano quel passaggio,

Presidente, colleghi, questo dibattito rischia seriamente di essere fuori tempo e fuori quadro. la dichiarazione, molto importante, del presidente degli Stati Uniti Obama chiarisce finalmente, dopo una lunga elaborazione ed esitazione, la posizione del nostro principale alleato e ci responsabilizza. Credo dunque, onorevoli

a confronto dei 160.000 presenti in Iraq nel momento di maggiore presenza militare. Dunque, ha marcato la discontinuità fondamentale dell'amministrazione americana: la fuoriuscita dall'Iraq e una diversa qualità militare e civile dell'impegno strategico della coalizione presente in Afghanistan.

la necessità di confermare o cancellare l'obbligazione internazionale dell'Italia. Io sono tra quanti, trovandomi all'opposizione al momento della decisione susseguente all'attentato

Non è il primo a farlo perché nella passata legislatura le forze della sinistra radicale hanno costantemente tenuto sotto scacco il Governo, di cui mi sono onorato di fare parte, proprio sulle missioni internazionali.

Bossi lo ha detto, ma non lo ha formalizzato: ha manifestato un malessere tradizionalmente obliquo da parte della Lega,

Voi siete andati a sostegno di Milosevic, esattamente come la sinistra estrema del nostro Paese! *(Applausi dal Gruppo PD).* Le forze democratiche, invece, avevano ben chiara in quella situazione drammatica da che parte si dovesse stare. io esprimo la posizione di chi ha ben chiaro da che parte si debba stare, e lo dico ai colleghi che hanno fatto parte della coalizione di centrosinistra così come a coloro che oggi responsabilmente come certamente farà la Lega - voteranno a favore di questo provvedimento ma irresponsabilmente davanti all'opinione pubblica immaginano di cavalcare questo malessere. Non è il momento di proporre il ritiro dei militari italiani dall'Afghanistan, gentile Presidente; non è il momento di proporre il ritiro dal Libano, dove l'Italia è richiesta e ha una funzione fondamentale; non è il momento di derubricare le di derubricare le nostre responsabilità nei Balcani, dove ci sono dei progressi ma ancora e tuttora delle criticità. È il momento di confermare la posizione che l'Italia ha avuto finora, e vorrei che questa fosse e restasse una posizione *bipartisan*,

esprimono linee dissenzienti. Questo è un fatto notevole. Quanto è avvenuto oggi con la presentazione da parte dell'Italia di un emendamento che chiede il ritiro entro febbraio del contingente italiano, non è un qualcosa che si possa affrontare come se fosse una dichiarazione domenicale alle agenzie di stampa, colleghi dell'Italia dei Valori: è una presa di posizione di un'estrema gravità. Un Governo, una maggioranza politica, una coalizione politica di maggioranza o di opposizione possono dividersi su una baruffa,

rappresenta una rottura politica, una discontinuità politica, che certo avrete assunto in maniera responsabile. Il collega Marcenaro giustamente è intervenuto

signor Presidente, la mia dichiarazione di voto favorevole a questo provvedimento, dentro la cornice che ho indicato: si tratta di un provvedimento assolutamente inaccettabile, non solo deludente per quanto riguarda la cooperazione

e in particolare di quella in Afghanistan, che è radicalmente condizionato dalla decisione presa dagli Stati Uniti. Perché è stata una decisione americana, ed è un fatto importante e sensibile. L'America ha deciso;

al termine di alcuni mesi di dibattito e di elaborazione che lo ha portato a scegliere in modo condizionato la richiesta del generale McChrystal, rappresenta una posizione che ci interpella; e qui noi dobbiamo decidere. Rompiamo le nostre alleanze internazionali? Cancelliamo unilateralmente, come ci propone l'Italia dei Valori, la nostra partecipazione ad una missione nella quale abbiamo avuto una funzione determinante fin dall'inizio, con sacrificio di uomini di risorse e di grande valore anche simbolico per il nostro Paese? Anche perché si deve rimettere in questione - su questo sono d'accordo - la natura e la qualità della strategia per sconfiggere Al Qaeda e per stabilizzare la situazione non solo in Afghanistan ma anche in Pakistan, poiché più che mai è chiara all'amministrazione americana l'unicità della questione. Non a caso, Obama fa riferimento ripetuto all'arsenale atomico del Pakistan e alla necessità di garantirne la messa in sicurezza come ad una delle missioni fondamentali, oltre all'operazione che è in corso da tempo da parte dell'esercito pakistano nelle aree occidentali del Paese confinanti con l'Afghanistan; il collega senatore generale Del Vecchio sa bene di cosa parliamo.

è indispensabile un processo di integrazione istituzionale e civile e di stabilizzazione delle istituzioni locali, al di là del momento elettivo presidenziale il cui svolgimento ben conosciamo. La posizione italiana assume oggi un maggiore valore

piuttosto, quella di contribuire - con le nostre forze, i nostri talenti e le nostre capacità, pur nelle condizioni ridotte di bilancio con le quali ci misuriamo oggi - a una definizione della strategia che permetta non una *exit una strategia di uscita, bensì una *success strategy*, ovvero una strategia di riuscita, in una missione che è interesse della comunità internazionale far sì che

su un'aliquota dell'IRAP, ma sulla politica estera. E oggi quello che è avvenuto somiglia molto da vicino alla rottura di un rapporto politico con l'Italia dei Valori.

non solo perché l'impegno del nostro Paese nelle missioni che garantiscono la pace nel mondo è un aspetto importante e qualificante dell'azione internazionale dell'Italia e non solo perché si tratta di un impegno ormai tradizionale, radicato, professionalizzato ed utile in tantissime parti del mondo. a favore di questo provvedimento anche e soprattutto perché vogliamo dare una testimonianza di serietà, di responsabilità e di sostegno ai nostri soldati che quotidianamente all'estero rappresentano il nostro Paese in situazioni di conflitto e in situazioni di particolare difficoltà e che meritano da parte del Parlamento uno sforzo comune, un sostegno e una solidarietà sincera, scevra da ogni forma di tatticismo. È stato già ricordato che l'Italia partecipa a 31 missioni a carattere multinazionale che operano sotto l'egida dell'ONU, dell'Unione europea e della NATO e, tra queste, le più impegnative sono quelle in Libano, in Afghanistan e nei Balcani. È chiaro che il tema è certamente politico; esso riguarda il ruolo che le forze politiche devono svolgere nel nostro Paese.

implicano sacrifici come quelli che i nostri soldati, anche in termini di vite umane, hanno fatto e stanno facendo nel mondo. Tutto questo non può tuttavia esimerci dal fare qualche considerazione di carattere critico, perché è evidente che anche gli eventi di questi ultimi giorni - mi riferisco, in particolar modo, all'Afghanistan - interrogano e devono interrogare il Paese, il Parlamento ed il Governo sulla strategia e sul cambio eventuale di strategia che l'Italia deve assumere. assumere. Alcuni rilievi di carattere critico sono importanti e fondamentali a partire dalla circostanza che nell'ultimo anno le modalità di finanziamento delle nostre missioni hanno perduto carattere di stabilità e certezza, che erano state assicurate a partire dall'istituzione dell'apposito Fondo missioni del 2003. Si è ridotto il periodo di copertura finanziaria delle missioni stesse da sei a quattro mesi e, infine, a due mesi nell'ultimo decreto o addirittura non è stato reiterato il finanziamento del Fondo speciale missione annuale nella finanziaria per il 2010. A questo riguardo, mi permetto di segnalare sommessamente che credo non sarebbe utile immaginare che a copertura del finanziamento e della ulteriore proroga che saremo chiamati a dare delle missioni internazionali del nostro Paese, queste vengano coperte *una tantum* con il gettito dello scudo fiscale. Mi sembrerebbe un modo non solo poco elegante, ma assolutamente politicamente e istituzionalmente inopportuno per sostenere uno sforzo internazionale del nostro Paese, che ha il carattere della stabilità e deve trovare nel bilancio dello Stato la stessa stabilità e la stessa certezza che intendiamo dare, con il nostro voto, alle missioni e ai militari impegnati all'estero. L'altra considerazione che mi permetto di svolgere è la seguente. È chiaro che, ad oggi, il cambio di strategia degli americani in Afghanistan, l'idea di una scansione temporale che preveda, in un primo momento, una forte implementazione delle risorse militari ed umane in quel Paese e, in un secondo momento, un'uscita da quel Paese impone anche a noi, (che di quella missione siamo stati e siamo ovviamente con ruoli diversi) di capire che cosa bisogna fare. E noi diciamo subito, con estrema chiarezza, che siamo favorevoli all'utilizzo di altri militari in Afghanistan: queste sono cose che vanno dette subito e con chiarezza. pretendiamo che il Governo venga in Parlamento e, a fronte delle novità che vengono dagli Stati Uniti, informi il Parlamento ed il Paese di quale sarà la strategia che intenderà utilizzare nelle varie missioni internazionali ed in particolar modo in Afghanistan, non solo sotto il profilo dell'impiego qualitativo e quantitativo degli uomini e delle risorse, e quindi anche di ciò che mette a disposizione per questo fronte comune di collaborazione futura; ma soprattutto per comprendere se e in che termini sia ancora valido ed attuale quel tipo di permanenza

del ruolo del nostro Paese in fronti come l'Afghanistan, evoca il ritiro o sollecita polemiche, tiene un atteggiamento irresponsabile indipendentemente dal merito della questione. Tiene un atteggiamento irresponsabile perché, in questo momento, ciò che tiene i nostri soldati lì, con uno spirito vivo, attento e presente è soprattutto il sostegno dell'intero Paese, delle istituzioni tutte e del Parlamento tutto; pertanto l'idea di dividersi, anche per una convenienza politica tutta interna, su un tema così importante, che qualifica l'identità, la presenza e lo sviluppo dell'attività del nostro Paese in quei terrificanti scenari di guerra, dove i nostri militari danno un supporto difficile, che diventa sempre più difficile di giorno in giorno, significa assumersi una responsabilità negativa, significa essere degli irresponsabili. Tutto ciò va stigmatizzato e prendiamo atto con favore che su questo tema vi sia anche da parte del Partito Democratico una posizione diversa, di assoluta responsabilità. Altrettanto attendiamo sul fronte della maggioranza, perché non si può andare nelle piazze e dire una cosa e poi venire in Parlamento e dirne un'altra: se sul tema delle missioni ci sono diversità di vedute nell'ambito del Governo e della maggioranza, ognuno deve assumersi la propria responsabilità, senza immaginare di agitare le piazze e poi fare discorsi diversi in Parlamento. Sul tema delle missioni internazionali dobbiamo lavorare per avere l'unità totale: l'unanimità del Parlamento è un sostegno forte che credo i nostri militari meritino e meriti ancora di più la vocazione che il nostro Paese ha dimostrato in questi anni in tutti gli scenari di guerra più difficili in cui è stato chiamato a collaborare.

Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il decreto-legge di proroga al 31 dicembre delle missioni militari in corso all'estero, varato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre scorso, giunge all'esame di questa Assemblea quando all'orizzonte si profila forse già la necessità di un'ulteriore proroga, almeno fino alla prossima estate.

Certamente da stanotte sappiamo che qualcosa è cambiato e che il Governo sarà in grado di spiegarci in modo esaustivo come conta di rispondere alle richieste che provengono da Washington. Ma è di altro che ora dobbiamo discutere. È importante comprendere che il nostro impegno militare è uno degli elementi a mio avviso fondamentali per incidere sulle dinamiche della politica estera.

peraltro in un contesto di crisi internazionale che sta attanagliando quasi tutti i Paesi. Dobbiamo decidere se convertire in legge questo decreto

che erano stati impiegati ad Herat per la gestione delle elezioni amministrative. Ricordo, inoltre, che - come è stato detto

sulla situazione geostrategica mondiale e, come hanno detto ieri alcuni colleghi, nel caso specifico il presidente Cantoni, di fronte a queste nuove sfide l'intera comunità internazionale è chiamata a svolgere un ruolo attivo, perché il mantenimento della pace e della sicurezza non può essere appannaggio

atto. È giusto ricordare poi che le nostre Forze armate hanno risposto sempre con grande coraggio, senso del dovere, professionalità e capacità operativa, qualità che pochi facendo guadagnare continuamente a noi parlamentari e al nostro Paese un significativo prestigio - non dobbiamo dimenticarlo - a livello internazionale ed un apprezzamento unanime da parte di tutti i consessi mondiali.

militari. Peraltro, le missioni internazionali, alla luce di questi fatti, si sono rivelate uno strumento assolutamente straordinario per tenere alto il nome del nostro Paese soprattutto all'estero

voglio precisare un'ultima cosa. Non possiamo dimenticare che durante l'approvazione di questo provvedimento, ancora una volta, qualcuno ha tentato di approfittare di questa occasione

in questo contesto. La Lega Nord, così come sempre ha fatto in passato nelle altre legislature, non può che aderire convintamente a questo provvedimento, perché convinta che è giusto portare a casa un risultato,

a trovare le condizioni per venire via da un Paese come quello non sconfitti, com'è successo ai russi. Sono convinto che i nostri Paesi siano importanti, che sanno ragionare e che porteranno a casa il risultato;

conferma una posizione che per noi è diventata una posizione di principio oltre che una posizione politica, quella che ci vede consapevoli delle responsabilità dell'Italia, nella proporzione e nella misura delle sue forze, nelle decisioni che la comunità internazionale assume e in quegli impegni che rientrano nel quadro del rispetto del diritto internazionale e di un concorso multilaterale della comunità internazionale. È un punto molto importante (non tornerò su una questione che ho sollevato in precedenza nel dibattito) per riaffermare quello che anche il collega Rutelli ha sottolineato, cioè che si tratta di un aspetto politicamente decisivo nella formazione degli orientamenti e degli schieramenti politici. Vorrei sottolineare questo impegno del nostro Paese si configura ormai da tempo - e dovremmo esserne più consapevoli - come un impegno strutturale, che non dipende solo dalle dalle singole missioni delle quali stiamo discutendo; è un impegno costante che nel mondo di oggi, nel mondo globalizzato, si richiede a tutti i Paesi per contribuire a per contribuire a realizzare quegli elementi di governo della situazione senza i quali il mondo sarebbe peggiore di quello che oggi conosciamo.

delle decisioni che oggi stiamo prendendo, dobbiamo sapere che forse affronteremo nei prossimi mesi, nel prossimo periodo, delle prove difficili e che in un conflitto come questo c'è bisogno anche c'è bisogno anche di una sostenibilità nei confronti di un'opinione pubblica che sia cosciente della natura dell'impegno che oggi prendiamo, del motivo per cui tante risorse che potrebbero essere attribuite ad altro sono destinate a questo impegno

Craxi, erano finanziate dal fondo imprevisti. Non possiamo ritornare al fondo imprevisti; c'è bisogno di costruire una dimensione permanente del nostro impegno e quindi anche una struttura del finanziamento

Quando si è consapevoli di questo impegno, abbiamo anche naturalmente bisogno di combinarlo con una responsabilità politica: la prima responsabilità, forse anche morale, è quella di essere capaci di contribuire con un'analisi realistica della situazione. Oggi un'analisi realistica della situazione di difficoltà, in cui in particolare nello scenario afgano le forze della coalizione internazionale si trovano, è un dovere: dobbiamo sapere come l'Italia anche

come cosa burocratica che prima o poi bisogna fare. Potete ricavare dal dibattito e dal confronto in Parlamento idee, proposte e forza.

se ne rendesse conto e provasse a valorizzare questo aspetto, farebbe cosa giusta. Siamo in una situazione molto difficile. Non commenterò il discorso che ha fatto a West Point questa notte il Presidente degli Stati Uniti, ma è evidente che parte dal riconoscimento di una sconfitta, di un arretramento. Obama parla di una sconfitta non irrimediabile, di una situazione non compromessa, ma naturalmente di questo parla. Aspettavamo le elezioni in Afghanistan come un punto di ripresa e sono state, invece, un punto di crisi:

di Negroponte, l'idea e l'ideologia dell'esportazione della democrazia secondo un modello solo ci ha portato a quel punto ed a quelle condizioni, invece che provare a trovare quelle soluzioni costituzionali adatte a quel Paese! Ma quanti errori di questo tipo sono stati stati compiuti! Vedi l'idea che fosse possibile una soluzione puramente militare e che la politica venisse in secondo piano. Oggi ho letto che il Presidente Obama dice: «Basta assegni in bianco a Karzai». Ma non si può pensare di investire sulla politica e di avere poi dall'altra parte un Governo di corruzione, di trafficanti. Su questo c'è una responsabilità che riguarda, secondo me, non solo la coalizione

mi chiedo perché il Governo è così reticente nell'affrontare una discussione politica e perché non fa fronte all'insieme dei suoi impegni. Lo ricordava il collega Rutelli: c'è una contraddizione tra la decisione che prendiamo oggi col voto della grandissima maggioranza del Parlamento ed il taglio che viene fatto ai fondi per lo sviluppo e la cooperazione, cioè dell'altra gamba, che andrebbe invece valorizzata, delle politiche da condurre. Questo è il punto il punto politico. Poiché stiamo discutendo di un provvedimento che riguarda una proroga di due mesi e, come qualcuno ha ricordato, il 28 gennaio ci sarà un appuntamento molto importante per quanto riguarda l'Afghanistan, poiché siamo in presenza di novità strategiche, come quelle annunciate dal Presidente degli Stati Uniti in queste settimane, vi chiediamo che di qua alle prossime settimane si ritorni su questo punto per organizzare in Parlamento una discussione politica sugli indirizzi, sulle scelte di fondo, perché anche su questo il Parlamento sia un punto di confronto, di discussione e di elaborazione. E ripeto: ripensate alla questione del fondo! Nessuno dice che non darete i soldi per le missioni internazionali; è una interpretazione meramente propagandistica e di poco conto. Non è questo il punto. Il punto è se, da un lato, si ha una visione di lungo periodo e, dall'altro, naturalmente se mettiamo questo aspetto un po' al riparo dalle oscillazioni contingenti della politica economica e se ci diamo atto fra noi che sono ancora il Ministero degli esteri e quello della difesa che decidono delle missioni internazionali e non il Ministero dell'economia, per quante buone ragioni possa avere! Non possiamo decidere di restare in Libano, in Afghanistan o in Kosovo sulla base dei conti di Tremonti - per quanto rispettabili essi siano lo dobbiamo decidere sulla base delle responsabilità che abbiamo. Questo è il punto. Non credo di dover aggiungere altro, se non il fatto che su fatto che su questo vorremmo una reciprocità, non del Governo o della maggioranza verso l'opposizione che non fa altro che esprimere con questo voto la sua convinzione di fare il proprio dovere verso il Paese; una reciprocità verso il Parlamento, considerato su questa come su altre questioni non una palla al piede, ma la sede che può anche per i nostri militari impegnati in situazioni così difficili e per il Paese al quale ci rivolgiamo un punto di riferimento più sicuro e unitario.

*(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando e che è stato analiticamente esaminato dalle Commissioni riunite esteri e difesa, che ho presieduto insieme al presidente Cantoni, e che è stato illustrato dai relatori, è essenzialmente volto a garantire la prosecuzione, per gli ultimi due mesi dell'anno, della partecipazione italiana alle missioni internazionali. Missioni autorizzate per il primo semestre dell'anno da un decreto-legge e per i successivi quattro mesi da una legge che le Commissioni esteri e difesa, della Camera prima e del Senato poi, hanno approvato con un voto unanime. Questa convergente volontà delle forze politiche è stata fino ad oggi il segno visibile dell'unità del Parlamento dietro la scelta di garantire un contributo importante, e in alcuni casi decisivo, alle missioni internazionali volte a garantire la pace e la stabilità in tanti importanti scenari. Sono tutte missioni decise e organizzate sotto l'egida delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali: la Nato e l'Unione europea in primo luogo. Dalla capacità di essere presenti nei più diversi scenari e di dare un contributo essenziale e apprezzato discende tanta parte del ruolo che l'Italia oggi svolge, e sempre più è chiamata a svolgere, sulla scena internazionale. È un'esperienza oramai quasi ventennale che ha visto l'Italia partecipare attivamente al mantenimento della pace e alla soluzione di crisi internazionali in coerenza con i principi fissati nell'articolo 11 della nostra Carta costituzionale. Governi di diverso colore hanno deciso la partecipazione dell'Italia a questa e a quella missione. E a esse non è mai mancato un ampio e trasversale sostegno parlamentare, che è la dimostrazione di una coerente e condivisa visione dell'Italia nel mondo. Col provvedimento che oggi approviamo, completiamo, prolungandola fino alla fine dell'anno, quell'autorizzazione politica e finanziaria a partecipare alle missioni che fu oggetto di una legge di iniziativa parlamentare *bipartisan* esaminata, come accennato, in sede deliberante dalle Commissioni riunite prima della pausa estiva. Ricordo che l'autorizzazione alla prosecuzione della nostra partecipazione alle missioni era stata introdotta nel decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, recante «provvedimenti anticrisi». Su iniziativa dell'opposizione e per volontà condivisa della maggioranza parlamentare queste norme furono scorporate da quel decreto e trasfuse in una autonoma iniziativa legislativa proprio per permettere su di esse un voto *bipartisan*, che fosse il segno visibile del sostegno dell'intero Parlamento nei confronti dell'azione dei nostri soldati, dei diplomatici e dell'altro personale impegnato nelle missioni.

Al di là dell'alternarsi dei Governi e delle maggioranze, occorre essere consapevoli, oggi più che mai, che la partecipazione alle missioni è un indispensabile elemento della politica estera del Paese. L'Italia è, e continuerà ad essere, un membro autorevole delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della NATO e un partner ascoltato dai suoi alleati se continuerà a dare un contributo qualificato e prezioso a queste missioni.

che la nostra Costituzione pone come obiettivo essenziale della partecipazione dell'Italia alla comunità internazionale e alle organizzazioni che ne costituiscono l'ordinamento. Come ben si capisce dal provvedimento che stiamo esaminando, l'Italia è impegnata in un consistente numero di Paesi; crescente è l'importanza della componente civile; gran parte delle risorse umane e materiali sono concentrate nelle missioni in Afghanistan, in Libano e nei Balcani. Queste ultime due sono tradizionali priorità strategiche del nostro Paese, che ha storicamente svolto un ruolo attivo e impegnato per la pace nei Balcani e nel Mediterraneo. La missione in Afghanistan è un importante contributo che noi diamo all'azione dell'Alleanza Atlantica, impegnata in uno scenario complesso e difficile al di fuori della sua tradizionale area di intervento. È in corso un'ampia riflessione sulla ridefinizione del concetto strategico dell'Alleanza, sul suo ruolo dopo la conclusione della Guerra fredda e la fine del cosiddetto secolo breve. La NATO, sempre più, deve essere uno strumento al servizio della legalità internazionale che vede nell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua fonte essenziale e il luogo naturale di confronto fra le nazioni. Con convinzione, la nuova amministrazione americana ha mostrato e mostra di voler operare in un quadro di relazioni multilaterali, rilanciando il ruolo delle Nazioni Unite, rafforzandone l'autorevolezza e la capacità di risolvere conflitti. L'Italia non dovrà mancare di dare il suo contributo per un rafforzamento della presenza internazionale in Afghanistan, dove è in gioco la nostra sicurezza e la credibilità stessa dell'Alleanza atlantica. Il Governo ci dirà quali saranno i termini del nostro ulteriore contributo. Più in generale, Più in generale, credo che l'Unione europea debba, in questo momento cruciale, rafforzare e strutturare ancor più la cooperazione transatlantica. Come ha chiaramente detto il presidente Obama, gli Stati Uniti sono consapevoli di non poter risolvere da soli i problemi proposti dall'agenda internazionale. Sempre più forte è l'esigenza di una responsabilità condivisa, di un rafforzamento dei fori multilaterali e delle organizzazioni internazionali. In questo quadro, nuove sfide si pongono all'Unione europea. Ieri è entrato in vigore il Trattato di Lisbona; con esso, l'Europa si dota di nuovi strumenti per svolgere, se ne avrà la volontà politica, un'autorevole azione sulla scena internazionale. Non posso nascondere una certa delusione per le nomine del nuovo Presidente del Consiglio europeo e, soprattutto, del nuovo Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. Tuttavia, dobbiamo impegnarci tutti perché queste nuove figure abbiano il sostegno politico e acquistino l'autorevolezza necessaria per poter proiettare efficacemente la voce dell'Europa nel mondo. Più in particolare, seppur resta per le decisioni di politica estera e di difesa il vincolo dell'unanimità, il Trattato di Lisbona prevede, per quest'ultima materia, una cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri che rispondano a criteri più elevati in termini di capacità militari e che abbiano la volontà politica di sottoscrivere impegni più vincolanti. Molte, già oggi, e in diversi teatri, sono le missioni civili e militari dell'Unione europea autorizzate e finanziate anche da questo decreto. Il futuro proporrà nuovi e più ambiziosi impegni. L'Italia dovrà partecipare sin dall'inizio a questa cooperazione strutturata, come partecipò sin dall'inizio all'Unione economica e monetaria. Ciò richiederà nuovi impegni e una ristrutturazione del nostro strumento militare. che ciò di cui discutiamo oggi - il finanziamento e l'autorizzazione a partecipare a missioni di pace - è oramai una funzione permanente e stabile della nostra politica estera, come anche della nostra politica di difesa. Signor Presidente, colleghi, riferendomi ad alcune affermazioni e richieste presentate da diversi senatori di maggioranza ed opposizione, ricordo che nelle Commissioni esteri e difesa della Camera dei deputati è in corso una riflessione, in parte già avviata nella scorsa legislatura, per elaborare uno strumento normativo che fornisca un quadro stabile a questo complesso di missioni. Un quadro che sia stabile quanto ai riferimenti normativi e alla disciplina da applicare al personale in missione, oltre che alle risorse finanziare da dedicare. È evidente come quest'ultimo aspetto, in una fase tanto delicata della nostra finanza pubblica, richiede interventi coraggiosi e un intelligente spirito riformatore. Sono sicuro che il Governo continuerà ad impegnarsi in quest'attività e auspico che la Camera dei deputati sappia proporre quanto prima al Senato un disegno di legge quadro sulla materia delle missioni, convincente e condiviso. Dall'efficacia e affabilità con cui riusciremo a rispondere alle richieste della comunità internazionale, e in particolare delle organizzazioni internazionali cui apparteniamo, dipendono, come accennavamo, gran parte del ruolo e del peso che il nostro Paese potrà continuare ad avere internazionalmente. Con questa consapevolezza e questo impegno dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà sul disegno di legge di conversione del decreto che stiamo esaminando. *(Applausi dal Gruppo PdL. Grazie non perché abbia trovato qualcosa con cui non potessi essere d'accordo nella dichiarazione di voto del senatore Marcenaro, né tanto meno con le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti d'America, il più citato nel nostro dibattito, il che la dice lunga su quanto invece ci sia da dire o da ascoltare da parte del Governo italiano.

prendere un'iniziativa di carattere diametralmente opposto rispetto ai fallimenti del proibizionismo e avviare, come era stato fatto nella scorsa legislatura, una serie di progetti che potessero convertire il papavero in morfina, per farne analgesici per quell'80 per cento del mondo che non li conosce. Il Governo italiano, più volte sollecitato, è rimasto silente né tanto meno ha voluto sondare eventuali altri Paesi europei in questa direzione. Il Governo italiano ritiene che, come si stia oggi in Afghanistan, sia il modo con cui dovremo continuare a restarci. Credo sia un problema da tenere in considerazione.

Grazie alla partecipazione di oltre 150 colleghi, a Ferragosto abbiamo visitato tutti gli istituti di pena presenti nel nostro Paese, rilevando

La situazione resta sicuramente al di fuori della Costituzione, ma altrettanto sicuramente al di fuori delle priorità di questo Governo.

ripeto ancora una volta - abbiamo visitato gli istituti di pena italiani, rilevando situazioni al di fuori della Costituzione e credo anche al di fuori della convivenza civile, seppure in un ambito ristretto, dove gli individui vengono privati della loro libertà e anche della loro dignità.

e di spendere almeno una o due ore il prossimo fine settimana per visitare le carceri della propria circoscrizione o collegio, anche perché in una dozzina di questi istituti sono in corso attività di protesta, di lotta non violenta,

per il rogo costato la vita a sette operai, contemporaneamente nello stabilimento di Terni è accaduto un altro incidente mortale: Diego Diego Bianchina, di 31 anni, addetto ai servizi ausiliari, ha respirato le esalazioni tossiche di acido cloridrico che stava travasando con un tubo da un serbatoio in alcune taniche. Desidero esprimere, come Italia dei Valori, il nostro cordoglio alla famiglia della vittima e la nostra solidarietà agli operai che ieri stesso hanno proclamato uno sciopero istantaneo di due ore, riversandosi sulle strade e chiedendo più sicurezza. Infatti, signor Presidente, siamo di fronte a condizioni di sicurezza davvero inaccettabili! Purtroppo, il risparmio è ancora oggi il primo obiettivo

il quale prevedeva ammende molto più pesanti per le imprese che non rispettano le norme di prevenzione e di sicurezza. Di fronte alle innumerevoli morti cosiddette bianche, è davvero raccapricciante pensare all'impatto che potrebbe avere

Mentre il Comune di Milano incamerava una perdita di 100 milioni di euro sui prodotti derivati, i manager di Unicredit festeggiavano per avere incassato un profitto di 2.040.000 euro in pochissime ore.

non rispondono: qualche giorno fa, nell'ambito di un'indagine conoscitiva sui prodotti derivati, sono stati auditi in 6a Commissione permanente i dirigenti di Unicredit

Davide Mereghetti e Luca Fornoni - hanno guadagnato un corrispettivo di 3,4 milioni di euro a testa, compensi calibrati su derivati truffaldini, e ho chiesto loro se il presidente Profumo avesse inviato una lettera di richiamo, una sanzione, li avesse licenziati, per fare in modo che queste persone non possano più nuocere, se stanno in banca con il mandato che viene loro dal presidente di Unicredit di piazzare prodotti truffaldini. Ebbene questi signori, manager di Unicredit, si sono rifiutati di rispondere alla mia precisa domanda. Colgo allora ancora una volta l'occasione - non sarà l'ultima - per sollecitare almeno la risposta

Presidente, torno ad affrontare il tema della FIAT di Termini Imerese. Come lei ben sa c'è stata un'apertura - a mio avviso timida e incompleta - da parte del Governo e una rigida posizione di risposta da parte della FIAT. della FIAT. Torno ancora una volta a porre una questione di metodo e di contenuto. Penso che di fronte ad una vicenda così importante, come è quella del futuro del settore dell'automobile in Italia,

incentivi. I Governi addirittura sono entrati direttamente nel merito dei piani industriali. Nello stesso tempo, signor Presidente, i Parlamenti si sono interessati e sono stati coinvolti direttamente

Produciamo poco rispetto al mercato interno e poco rispetto al mercato internazionale. E allora, signor Presidente, è necessario che questa vicenda strategica, di vitale importanza per l'assetto industriale del nostro Paese, trovi spazio solenne in Parlamento. Lei sa che i lavoratori e le organizzazioni sindacali sono giustamente preoccupati. Già ci sono delle prime iniziative spontanee. Il Parlamento non può essere tagliato fuori. Deve dare voce e rappresentanza

di Termini Imerese è incompleta, ma c'è un'opera che è vitale e decisiva per le sorti dello stabilimento FIAT ed è il porto, che è già pronto;

che si potrebbe facilmente raggiungere anche con un collegamento diretto dallo stabilimento. L'altro fatto, Presidente, sono gli incentivi messi a disposizione dalla Regione. Non c'è alcuna Regione d'Italia, dove c'è uno stabilimento, in cui non si sono messi sul tappeto della negoziazione e delle convenienze una tale massa di opportunità, interessanti perché puntano sull'innovazione e perché creano le condizioni per un grande rilancio della FIAT in Sicilia, a Termini Imerese. Ecco perché torno a chiederle una discussione parlamentare, una comunicazione da parte del Ministro delle attività produttive qui in Parlamento in modo che il Parlamento sia coinvolto in modo solenne e diretto. Signor Presidente, è vitale farlo ed è bene che sia fatto adesso, perché ancora la negoziazione aperta, è bene che si intervenga prima che le proteste diventino roventi, è bene che il Parlamento dia al Governo quella forza che il Governo ancora non ha dimostrato di avere, che è quella di avere un tavolo dove far pesare il meccanismo degli incentivi. Tra l'altro, signor Presidente, preannuncio che aderirò alla richiesta che proviene dai lavoratori, dalle organizzazioni sindacali, dal comune, dalla Provincia e dalla Regione Sicilia, che è quella di chiedere ai parlamentari meridionali, in particolare siciliani, di non votare il meccanismo, seppur positivo, degli ecoincentivi che ancora una volta la FIAT torna a chiedere. Non possiamo infatti accettare un'idea, che è quella di ridimensionare la produzione di automobili in Italia e, ancora peggio, di ridimensionarla a partire dalla Sicilia: è una scelta sbagliata, rovinosa su cui penso il Parlamento debba intervenire facendo venire in Aula il Ministro delle attività produttive.

letto nel suo intervento quanto egli ha detto: «Signor Presidente, il problema della FIAT in Sicilia non può essere liquidato con un banale intervento, come quello fatto dal senatore Garraffa».

mio intervento e che riporto: «Oggi sia Marchionne che le televisioni pubbliche» - e, aggiungo, anche dirigenti della stessa FIAT - «hanno detto che il Governo regionale precedente doveva garantire determinate risorse».

La verità è che quelle opere non sono state compiute perché il Governo siciliano, per le vicissitudini vissute dal senatore Cuffaro, non è rimasto in carica. nel mio ruolo di Vice Presidente della Commissione industria, avendo su questo tema discusso ampiamente in Commissione anche per quanto riguarda l'Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco,

di ieri ha liquidato la vicenda FIAT di Termini Imerese in pochissimo tempo, con una innata subalternità nei confronti del dottor Marchionne, si presenti in Aula: ripeto, chiedo che il ministro Scajola venga in Aula, e lì gli chiariremo le idee.

per svolgere alcune precisazioni al fine di evitare che l'opinione pubblica venga orientata in modo non corretto rispetto alla vicenda della FIAT di Termini Imerese.

a mettersi a disposizione dello stabilimento FIAT di Termini creando un grande squilibrio nella produttività e negli investimenti dei medesimi imprenditori del settore.

La questione FIAT quindi non può rimanere fuori dalle Aule parlamentari. La questione FIAT non può rimanere fuori dall'attenzione di un Parlamento che deve necessariamente essere coinvolto da un problema che sta mettendo in ginocchio le scelte politiche e industriali di questo Governo nel Meridione d'Italia

Non serve continuare a investire soldi per fare contratti di programma, che non si possono fare semplicemente perché, essendo la FIAT una grande impresa, le

altri incentivi se la FIAT non prende l'impegno a tenere lo stabilimento di Termini Imerese aperto a fare macchine. Perché se dovesse fare bulloni, come afferma Marchionne, dal momento che vi

di valutare l'opportunità di invitare il Ministro a riferire in Aula sulla questione di Termini Imerese. Ovviamente, tocca a ciascuno di voi valutare l'opportunità di presentare una mozione per coinvolgere l'Aula del Senato in un dibattito approfondito su quella che non mi sembra una questione territoriale, ma una questione di carattere nazionale. Lascio, quindi, alle vostre valutazioni l'opportunità di far partecipare tutta l'Aula a questo dibattito. **Saluto ad una